Tra le altre cose, mi pare da sottolineare il fatto che la tecnica legislativa che adottiamo in questo caso sia quella preferibile, che auspicheremmo vedere normalmente. Se c'è una norma penale il cui ambito di applicazione non è chiarissimo, rispetto a un fatto che solleva un allarme sociale, anziché creare nuovi reati, come questa maggioranza fa al ritmo di uno al mese, nonostante le dichiarazioni avverse al panpenalismo,

migliorare l'ambito di applicazione della norma e di fare in modo che un fenomeno che crea allarme sociale sia indirizzato in modo appropriato non tanto per l'opinione pubblica, quanto verso la repressione del fenomeno criminale, che è quello che ci dovrebbe interessare di più. Mi sembra quindi un modo di operare corretto, anche se la norma in quanto tale, a mio avviso, mostra ancora qualche elemento di indeterminatezza, come ad esempio il riferimento generico all'età,

furono presentati nella scorsa legislatura anche alla Camera), merita sicuramente un percorso abbreviato, in quanto non avrebbe senso ricominciare da zero un percorso che il Senato nella scorsa legislatura aveva già concluso. Pertanto, senza ombra di dubbio e pur permanendo qualche perplessità sul merito della norma, il Gruppo Azione-ItaliaViva-RenewEurope voterà favorevolmente alla procedura abbreviata per questo disegno di legge.

Questo provvedimento interviene su un tema che quindi non può che essere particolarmente sentito. Molte di queste truffe hanno a che fare con finti fornitori di luce,

sono all'ordine del giorno persone che circolano spacciandosi per incaricati di gestori vari (ormai, con la liberalizzazione delle tariffe, sta accadendo anche questo) e che sostanzialmente convincono persone prive di difese, come può essere una persona anziana, minacciando chissà cosa. qualcuno è stato detto addirittura che per legge doveva cambiare le regole tariffarie del proprio contratto di fornitura di energia elettrica o gas; spesso vengono utilizzate addirittura informazioni sugli affetti più cari (figli, nipoti) per arraffare contanti e gioielli, per indurre una sorta di panico adducendo incidenti, guai con la giustizia o situazioni di pericolo. Si tratta, come dicevo, di comportamenti odiosi e di reati che aggiungono meschinità a comportamenti illegali.

Il codice penale, all'articolo 643, già punisce con la reclusione e con una sanzione pecuniaria chiunque per procurare per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o dell'inesperienza di una persona minore ovvero dello stato di infermità e deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induca a compiere un atto che comporti qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso. Le condizioni necessarie per la sussistenza del reato sono quindi rappresentate dall'esistenza di un'infermità o di deficienza psichica, la cui conoscenza da parte dell'autore costituisce premessa indispensabile. Non vi è alcun dubbio che l'anziano possa essere vittima privilegiata di questo genere di reato e i fatti di cronaca purtroppo lo dimostrano. La vulnerabilità specifica che caratterizza l'anziano lo espone difatti, in maniera particolare, al rischio di rimanere vittima di suggestioni, pressioni ambientali e influenze esterne; in altre parole, a quell'attività di induzione a compiere atti giuridici di per sé dannosi, che costituisce uno degli elementi fondanti del reato di circonvenzione. Possiamo quindi ritenere che l'introduzione di una norma specifica dedicata al requisito dell'anzianità sia una sorta di *alert* particolare, una lampadina che accendiamo e che, aggiungendo di fatto poco alla norma esistente, richiama l'attenzione del giudice su una particolare condizione, anche in riferimento all'età della vittima. Il provvedimento in discussione non rappresenta di certo una rivoluzione in ambito penale, quanto una sua più precisa definizione, andando a riempire in via legislativa una lacuna spesso già colmata dalle interpretazioni dei tribunali e dei giudici. Pertanto, la richiesta di adozione della procedura d'urgenza, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, che consente, entro sei mesi dall'inizio della legislatura, di riprendere i progetti di legge che non hanno avuto completamento, ci vede assolutamente favorevoli, non perché siamo giustizialisti - è ovvio - o perché pensiamo che soltanto la punizione sia sia l'elemento di soluzione a un problema, ma perché è vero che nel nostro ordinamento c'è una lacuna che può condurre all'impunità di chi ha commesso reati di truffa ai danni degli anziani. anziani. Per evitare che questo accada, siamo consapevoli che è necessario il voto favorevole sulla procedura d'urgenza di un provvedimento che deve giungere al termine. Con questo voto possiamo completare l'*iter*. Signor Presidente, anche Forza Italia voterà a favore della richiesta di procedura d'urgenza su questo provvedimento, che - com'è già stato ricordato dagli oratori che mi hanno preceduto - aveva già avuto il via libera da parte di questo Senato nel 2019. È un provvedimento che va a incidere, normare e dettagliare meglio una fattispecie di reato particolarmente odiosa, che vede come vittime soprattutto gli anziani. Da questo punto di vista, quanto riferito poc'anzi dalla collega Cucchi non può che essere sottoscritto, nel senso che la cronaca quotidiana ci mette in evidenza tutta una serie di truffe ai danni delle persone più vulnerabili e più fragili che sono gli anziani, addirittura spesso facendo leva su presunti e inesistenti drammi umani che hanno interessato i congiunti. Sotto questo profilo, la necessità di un provvedimento c'è. Io sono anche relatore in Commissione del testo e probabilmente - come diceva giustamente il collega Scalfarotto - sarà necessaria qualche incisione chirurgica

Signor Presidente, onorevoli colleghi, negli ultimi cinquant'anni l'invecchiamento della popolazione italiana è stato uno dei più rapidi tra i Paesi maggiormente sviluppati e si stima che nel 2050 la quota di ultrasessantacinquenni ammonterà al 35 per cento della popolazione totale, con un'attesa di vita media pari a 82,5 anni. Oggi gli *over* 65 in Italia sono 14 milioni e costituiscono il 23 per cento della popolazione, ma quanti sono gli anziani fragili? I dati provengono dal sistema di sorveglianza Passi d'argento dell'Istituto superiore di sanità, che ogni anno completa un ampio sondaggio fra campioni di popolazione. Nel periodo 2017-2020, il 18 per cento interrogati è considerato fragile, cioè bisognoso di assistenza: nel 93 per cento dei casi ricevono aiuto dai familiari, spesso altrettanto anziani,

Di recente, in quest'Aula abbiamo discusso il cosiddetto disegno di legge anziani, in vigore dal 31 marzo 2023. La norma in attuazione del PNRR avvia politiche in favore delle persone anziane, specie quelle non autosufficienti, con una nuova organizzazione assistenziale. Il MoVimento 5 Stelle ha contribuito ad apportare modifiche migliorative del testo, sebbene abbia rimarcato fortemente che l'assenza di risorse da destinare a questa riforma, così come la scarsa attenzione

Gli anziani vittime di truffa sono prevalentemente uomini tra i sessantacinque e gli ottant'anni, soglia oltre la quale le vittime di sesso femminile superano quelle di sesso maschile. Il truffatore trae in inganno la vittima attuando artifizi e raggiri, approfittando della sua buona fede e dell'ingenuità e facendo affidamento sulle eventuali ridotte capacità di reazione e di critica, nonché del suo bisogno di avere relazioni sociali. La categoria degli anziani è infatti caratterizzata da alcuni fattori di vulnerabilità, come l'età anagrafica, il minor vigore fisico e psicologico, in alcuni casi un livello di istruzione non elevato e, non ultimo, un forte bisogno di comunicare. centinaia di casi di truffe al mese. Ogni 100.000 abitanti si rilevano 402 anziani vittime di furto, 24 vittime di truffa e sette di rapina. Valori più elevati sono riscontrati in Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Toscana e Lazio. La situazione, secondo il giudice Alessandro Arturi, sta assumendo le connotazioni di una vera e propria emergenza sociale, destinata a suscitare un allarme diffuso nella popolazione e a tradursi in un senso generalizzato

le persone più deboli e indifese. In questa sede ci accingiamo ad esprimere il voto sulla richiesta di procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento come forza di opposizione, ci piacerebbe rafforzare con la stessa urgenza le tutele nei confronti dei fragili e degli anziani anche in termini di risorse e di fondi (neanche di recente il DEF ne ha appostati).

e interveniamo quando il reato è ormai stato commesso e l'anziano, il fragile, ha già subito il danno peggiore. Tuttavia, proprio per l'attenzione e la vicinanza alle persone fragili e agli anziani

è la riproposizione di un atto del Senato, il n. 980, che era già stato approvato nella scorsa legislatura, tra l'altro con il voto favorevole di tutti (se non ricordo male, ci fu solo un'astensione).

la persona che è stata truffata sostanzialmente versi in uno stato di incapacità o di minorazione della sfera intellettiva. Se invece ci si trova di fronte al caso di un anziano che è semplicemente in una condizione di vulnerabilità, le pene sono lievi e sostanzialmente chi truffa gli anziani la fa sempre franca. Questo è il motivo per cui sono in aumento questi reati nel nostro Paese, come tanti altri, perché comunque chi li commette alla fine non viene

colui che raggira una persona che si trova in uno stato di bisogno ovvero che abusa di una condizione di debolezza o di vulnerabilità, vulnerabilità, tipica di una persona anziana. In questo Paese, se vogliamo ripristinare l'ordine e la legalità, dobbiamo fare in modo che chi sbaglia paghi davvero

facciamo quello che vogliamo, tanto alla fine nessuno viene punito. Questo è il principio: poi, è giusto che siano fatte le dovute valutazioni e non bisogna mai estremizzare, né in un senso, né nell'altro; penso però che negli ultimi tempi si sia un po' troppo estremizzato nell'altro. Chi commette questi raggiri e queste truffe spesso, queste truffe spesso, anzi quasi sempre, resta impunito. Allora interveniamo come Parlamento. Visto che vogliamo fare prevenzione, cominciamo a far capire che chi sbaglia paga e vedrete che poi qualcuno la smetterà di raggirare e di truffare i nostri anziani. Questa è la logica che ispira il disegno di legge che è stato approvato da tutti, motivo per cui voteremo favorevolmente alla riproposizione, attraverso la procedura abbreviata, di questo provvedimento. Signora Presidente, anche il Gruppo Partito Democratico voterà a favore di questa proposta di urgenza e di accelerazione dell'*iter* procedurale del disegno di legge che riguarda le truffe nei confronti degli anziani. Voteremo a favore perché condividiamo lo spirito e la *ratio* della legge, che peraltro - com'è già stato ricordato - nella scorsa legislatura venne approvata pressoché all'unanimità dal Senato e poi non venne approvata definitivamente dalla Camera per problemi di ingorgo dei lavori in Commissione. Venne approvata all'unanimità perché

Il disegno di legge attrae alla fattispecie della circonvenzione di incapace condotte che oggi sono invece attratte dal reato di truffa. La circonvenzione di incapace punisce con pene

già nel recente passato, nella precedente legislatura. E bene hanno fatto a riproporlo, in questa legislatura, per cercare la convergenza di tutti quanti noi su un provvedimento del genere. Come diceva la senatrice Cucchi, che mi ha preceduto,

una riflessione portata in Commissione proprio ieri dal collega Scarpinato, il quale ha detto di provare a immaginare quattro energumeni che sfondano la porta di un anziano, gli entrano in casa, lo raggirano, lo derubano e magari lo maltrattano.

L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla richiesta di adozione della procedura abbreviata, prevista dall'articolo 81 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 551.

firma con un discorso alla Camera la sua condanna a morte. "Tempesta", come viene chiamato dai compagni di partito per il suo carattere battagliero, ne è consapevole, perché, appena finito di parlare, dopo aver denunciato pubblicamente l'uso sistematico della violenza a scopo intimidatorio usata dai fascisti per vincere le elezioni e contestato la validità del voto, dice ai colleghi: «Io il mio discorso l'ho fatto. Ora voi preparate

Pochi giorni dopo, il 10 giugno, viene rapito a Roma. Sono da poco passate le quattro del pomeriggio, una squadra di fascisti lo preleva con la forza e lo carica in auto, dove viene picchiato e accoltellato fino alla morte, per poi essere seppellito nel bosco della Quartarella, a 25 chilometri dalla Capitale. Il provvedimento di cui stiamo discutendo intende ricordare e celebrare nel 2024, a cento anni dal rapimento e dall'omicidio, la figura e il pensiero di Giacomo Matteotti,

quanto che sia necessaria la vera e propria formazione di una coscienza civile, come indispensabile avvio verso una più profonda comprensione dei processi dinamici attraverso i quali si svolge la vita dei popoli e si determina l'evoluzione delle diverse forme della vita associata. Ricordare Giacomo Matteotti, deputato, uomo politico e studioso che ha interpretato i sentimenti più alti dell'Italia e non ha voluto piegarsi alla dittatura nascente, vuole avere quindi soprattutto il significato di un monito a difesa della libertà e della democrazia, principi fondanti della Costituzione italiana. È molto importante infatti, soprattutto in un tempo storico come questo, promuovere il recupero della memoria e provare a sviluppare, specialmente nelle giovani generazioni, la consapevolezza storica e la coscienza del proprio ruolo sociale e dell'appartenenza alla comunità civile, ossia la capacità di distinguere le unità di informazione e le unità di giudizio nella ricostruzione dei fatti storici. Da questo punto di vista, consideriamo questo un provvedimento che può effettivamente rappresentare un'opportunità di scelta culturale, pedagogica e didattica per investire nella memoria

della figura storica di cui stiamo discutendo, Giacomo Matteotti, permettetemi di dire che un provvedimento per la sua celebrazione è fin troppo tardivo.

diventi effettivamente patrimonio della coscienza pubblica attraverso quello che è più importante, ossia la promozione, anche mediante l'assegnazione di apposite borse di studio *(Applausi)* rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado, della ricerca storica e dello studio avente ad oggetto la vita, il pensiero e l'opera di Giacomo Matteotti, con particolare riferimento alle sue attività in ambito sindacale, come amministratore locale, studioso e naturalmente parlamentare, nonché al periodo storico compreso tra la Prima guerra mondiale e la sua morte. Altrettanto importanti saranno naturalmente i contributi previsti, che verranno dalle istituzioni scolastiche. Insomma, con il provvedimento in esame ciascuno di noi potrà concorrere meglio e a divulgare la storia di questo glorioso martire d'Italia con la nobile volontà di far sapere la verità, ossia che negli ultimi cento anni di storia nazionale uomini come lui e figure come la sua

per essere stata promotrice di questo importante provvedimento, nonché per il suo impegno civile e politico, affinché la memoria di sangue che ha caratterizzato e attraversato il nostro Paese resti nella memoria collettiva per non essere dimenticata. Ringrazio altresì il senatore Verducci per il suo prezioso lavoro di relatore. del Governo, colleghi, il mio sarà un intervento molto breve, perché il Gruppo Per le Autonomie si riserva un intervento più compiuto in sede di discussione generale, quando arriverà in Aula il vero e proprio

Il secondo aspetto è quello che riguarda il ruolo che ha avuto l'Assemblea del Senato nel processo a carico di quelli che sono stati considerati i mandanti del delitto Matteotti. Gli archivi del Senato sono molto ricchi di materiale che varrebbe la pena di essere ripreso in considerazione del ruolo che la politica di allora ha avuto in tutta questa vicenda. Ci Ci auguriamo che l'*iter* legislativo proceda speditamente e si possa tornare presto in Aula per parlare del merito. C'è poi un aspetto territoriale che, come Gruppo Per le Autonomie, abbiamo ritenuto di sottolineare, ossia che i natali di Giacomo Matteotti sono nel territorio del Trentino. Per questo motivo ci auguriamo di procedere quanto prima all'esame di merito.

senatrice a vita Liliana Segre e al presidente dell'allora Commissione cultura, il collega Riccardo Nencini. Ringrazio altresì tutte le colleghe e i colleghi e anche l'attuale Presidente della Commissione cultura e il vice presidente presidente Versace. È un ringraziamento vero perché - com'è stato detto precedentemente dai colleghi quello di oggi non è soltanto un atto storico e parlamentare, ma è un patrimonio della nostra stessa identità nazionale. Celebrare i cento anni dalla morte di Matteotti, quindi, è un atto importante, perché significa ricordare un uomo che ha combattuto per la libertà. E dirlo oggi in quest'Aula, pochi giorni dopo il 25 aprile, pensando anche alle importanti celebrazioni nazionali che si svolgeranno nelle prossime settimane,

collega De Cristofaro - è importantissimo trasmettere questo valore e questi ideali soprattutto alle attuali e alle nuove generazioni. Ricordare chi ha combattuto per la libertà, ma in modo particolare Giacomo Matteotti, significa ricordare anche la prima vera reazione al fascismo, che vi fu il 27 giugno 1924, con la secessione dell'Aventino. La libertà, quindi, è un atto forte, che richiede coraggio e comporta rischi e grandi responsabilità. Matteotti era da solo era da solo e poi, man mano, fu accompagnato da pochi altri nella sua strada. Lo seguirono due liberali, entrambi poi uccisi, come Gobetti e Giovanni Amendola, padre di Giorgio Amendola, assieme a pochi socialriformisti, alla figura di don Sturzo e a una parte della sinistra, anche massimalista, che però non la pensava come lui.

considerato quasi un male in quel periodo storico e che anche oggi - e siamo nel 2023 - fa fatica ad affermarsi - fatemelo dire - proprio perché essere riformisti significa

richiamare quel pensiero e quel patrimonio ed essere tutti noi, senza distinzione di colore politico, classe dirigente del Paese. Paese. I riformisti devono riprendere il cammino della buona politica, perché - come ci insegna Matteotti - la politica senza etica e senza valori diventa mera gestione della cosa pubblica. Mai come in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo - dal punto di vista internazionale, dei conflitti e delle guerre civili, ma anche della grande crisi economica, sociale, culturale

e riflettere su quanto sia importante, oggi, vivere in un Paese libero e democratico. Lo dobbiamo a figure storiche fondamentali come quella di Giacomo Matteotti. il nostro vivere quotidiano e il nostro ruolo di parlamentari e di liberi cittadini devono essere attualizzati ogni giorno, ricordando figure come queste e facendo in modo che tale patrimonio diventi per noi fondamentale nell'azione politica quotidiana.

e chi ne ha una superficiale conoscenza lo ricorda solo come vittima di un efferato crimine, disconoscendone il pensiero e la cultura politica, che sono il tratto più affascinante. Quell'assassinio ha violentato non solo una persona e il suo patrimonio di umanità e di affetti, ma anche una più generale libertà di pensiero e di iniziativa politica, nonché il pluralismo e i diritti delle minoranze. Quando il dibattito politico si mescola con la protervia, la violenza e la sopraffazione, l'uomo ritorna alla preistoria e quell'evento fu una regressione della civiltà, unitamente ad altre barbarie che si consumarono, che ancora oggi occorre ricordare e su cui bisogna riflettere, senza andare alla ricerca del medesimo crimine di segno opposto, quasi a compensare le ferite subite con altri danni. È una modalità un po' infantile di giudicare le cose. Quando pensiamo a quello che è successo, ci sembra di stare in un'altra epoca. Se però leggiamo gli scritti di Matteotti, ne scopriamo il carattere di attualità e il senso di preoccupazione per quello che stava avvenendo e non possiamo certo dire che fosse la conseguenza di ignoranza diffusa, perché abbiamo la condivisione di grandi intellettuali, i manifesti. Penso a intellettuali del calibro di Giovanni Gentile, di Marinetti, di Pirandello, di Ungaretti e di Curzio Malaparte e anche a quelli più critici, come Benedetto Croce, che sottovalutarono gli eventi e votarono la fiducia al Governo anche dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti. Tutto questo è successo solo nel secolo scorso e anche oggi nel mondo assistiamo a sopraffazioni, prese di potere con invasioni, guerre e omicidi di Stato; miliardi di persone vivono sottoposte a dittature con Governi non democratici. La storia, si sa, è ciclica, come diceva persino Machiavelli: tutti i tempi tornano e gli uomini sono sempre i medesimi. Esiste solo la capacità dell'uomo di dominare il corso degli eventi, utilizzando opportunamente le esperienze degli errori compiuti nel passato, cioè le strade da non ripercorrere. Per chi reputa non opportuno richiamare la nostra radice cristiana, rapportandosi per esempio ai concetti di amore e di fraternità cristiani, basterebbe oggi giudicare obiettivamente le cose con il metodo dell'etica costituzionale. Oggi abbiamo questo grande criterio di giudizio, una preziosa bilancia attraverso la quale pesare gli uomini e la storia, come se fosse una chiave magica che apre tutte le porte della valutazione degli accadimenti ed è a disposizione di tutti. Anche nelle relazioni internazionali conflittuali, che rappresentano l'unico ambito in cui la Costituzione legittima l'uso della forza, lo fa in un'ottica difensiva e di protezione della propria integrità e giammai legittima la mera rabbiosa ritorsione finalizzata ad arrecare del male. In tal senso, ricordare Giacomo Matteotti ci serve in fondo a ricordare la Costituzione, di cui egli fu precursore con i suoi principi di socialismo riformista, oscurati dall'unica memoria dell'efferato omicidio. Il centenario dovrà servire soprattutto a questo: disvelare la portata storica del suo messaggio politico, stimolando iniziative che ripercorrano la sua vita, che, da figura di spessore nazionale all'ingresso a Montecitorio alla segreteria del Partito Socialista Unitario, racconta l'impegno nella lotta al fascismo, ma anche l'idea di politica come demagogia. La prima lezione che ci viene dalla vita e dalla morte di Giacomo Matteotti è perciò la difesa strenua della democrazia e la lotta per la sua continua evoluzione, tesa al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del popolo. La seconda lezione è la lotta contro la violenza e la sopraffazione come mezzi di conquista del potere. Vi è poi un'altra lezione, che riguarda il coraggio come virtù civile: Giacomo Matteotti sapeva benissimo a cosa andava incontro, eppure fece quel discorso;

La quarta lezione è la difesa della politica come servizio e progetto. In realtà, per Matteotti la politica era solo un pretesto: quello che contava erano gli uomini e la loro vita. Va ricordata la straordinaria mole di lavoro di formazione degli amministratori e dei sindacalisti. Bisogna recuperare il suo pensiero, che è stato di notevole spessore, ma che è finito quasi nell'oblio, oscurato dalla sua tragica fine. Noi siamo una coalizione democratica e di Governo - e finisco, signor Presidente - che non ha timore di misurarsi con i più preziosi principi costituzionali, avendo a cuore l'obiettivo di conciliare la cultura democratica e dei diritti sociali con quella liberale e del merito. Ci sentiamo quindi compartecipi di un'iniziativa legislativa, non solo per ricordare una rilevante ricorrenza storica, ma anche per promuovere la conoscenza della cultura democratica che, nelle varie articolazioni storicamente assunte, ha contribuito in maniera decisiva alla lotta contro il totalitarismo, a costruire la costituzione della Repubblica, a sviluppare la democrazia costituzionale

Signor Presidente, il disegno di legge n. 551 riproduce il testo approvato dal Senato il 19 maggio 2022 (Atto Senato 2317), rimasto pendente alla Camera dei deputati per la conclusione anticipata della legislatura. Il provvedimento ha come titolo «Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti» e intende ricordare e celebrare, a cent'anni dal rapimento e dall'omicidio, la figura e il pensiero del deputato socialista vittima della violenza fascista. Come ricorda la relazione illustrativa al disegno di legge, Matteotti non fu il primo e non sarà l'ultimo parlamentare - prima di lui Giuseppe Di Vagno e dopo di lui Giovanni Amendola - ad essere ucciso dallo squadrismo per aver difeso la sorte degli ultimi e la libertà. Eppure, risale proprio alla sua morte la trasformazione definitiva del regime, già illiberale, in autentica dittatura, dopo i lunghi mesi di difficoltà in cui il Governo Mussolini si era imbattuto. Al suo rapimento e omicidio, commessi il 10 giugno 1924, seguì la secessione dell'Aventino. Mesi dopo il ritrovamento del suo cadavere, avvenuto il 16 agosto, Mussolini, con un discorso a Montecitorio il 3 gennaio 1925, dichiarò conclusa la questione Matteotti e dispose la fine della libertà di stampa e l'emarginazione delle opposizioni. Questa è la data che viene indicata come spartiacque nella storia d'Italia, segnando l'inizio della dittatura. Ricordare Giacomo Matteotti, un deputato, un uomo politico e uno studioso che ha interpretato i sentimenti più alti dell'Italia e non ha voluto piegarsi alla dittatura nascente, vuole avere quindi soprattutto il significato di un monito a difendere la libertà e la democrazia sempre e comunque. L'articolo 1 del disegno di legge in questione prevede che le celebrazioni siano finalizzate a promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale. L'articolo 2, nel disciplinare le iniziative per il centenario della morte di Matteotti, statuisce che lo Stato riconosce meritevoli di sostegno e finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, delle opere, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla sua figura. Tali progetti Tali progetti possono essere realizzati anche in collaborazione con soggetti pubblici, associazioni, fondazioni e istituti culturali, attraverso iniziative che possono sostanziarsi in attività celebrative, convegni nazionali e internazionali, iniziative didattico-formative e culturali per promuovere in Italia e all'estero la conoscenza della vita, del pensiero e dell'opera di Giacomo Matteotti. Le iniziative in questione possono sostanziarsi nella promozione, anche mediante l'assegnazione di apposite borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado, della ricerca storica e dello studio aventi a oggetto la vita, il pensiero e l'opera di Matteotti, con particolare riferimento alle sue attività in ambito sindacale, come amministratore locale, studioso e parlamentare, nonché al periodo storico compreso tra la Prima guerra mondiale e la sua morte. nella raccolta, nella conservazione, nel restauro, nella manutenzione e nella digitalizzazione dei documenti relativi all'attività di Matteotti, nonché nella pubblicazione di materiali inediti e nella promozione di iniziative didattiche e formative, attraverso il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici e dell'intero territorio nazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione. L'articolo 4 prevede l'assegnazione alla Casa Museo Giacomo Matteotti di Fratta Polesine, suo luogo di nascita, di una particolare dotazione economica, non solo per la promozione di eventi, ma anche per sostenere interventi di manutenzione e restauro necessari alla fruizione pubblica del museo medesimo e per la raccolta, catalogazione e digitalizzazione di documenti relativi alla sua attività. Il nostro Gruppo, Presidente, crede che sia fondamentale la divulgazione del ricordo dell'opera e del pensiero di Giacomo Matteotti: se oggi noi tutti siamo qui abbiamo l'onore di rappresentare le istituzioni democratiche del nostro Paese, è anche grazie al lavoro, al pensiero e al sacrificio di Giacomo Matteotti. È per questo che annuncio il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

che di fatto celebra la ricorrenza del centenario dal rapimento e dall'omicidio di Giacomo Matteotti, noi non siamo d'accordo, siamo stra-d'accordo, e lo diciamo al presentatore, senatore Verducci.

si disposero la fine della libertà di stampa e l'emarginazione delle opposizioni e si andò verso il regime fascista.

rappresenta un monito a difendere libertà e democrazia sempre e comunque. difendere libertà e democrazia sempre e comunque. Permettetemi una piccola osservazione su quello che sta succedendo oggi, su chi sostanzialmente minaccia

costituiscono una minaccia esterna. Non dimentichiamo però che esiste anche una minaccia interna, che si chiama «politicamente corretto» o «pensiero unico e dominante» e sapete perché? Se si parla di libertà, dobbiamo parlare anche di questo.

sostiene che è giusto che tra Ucraina e Russia si raggiunga al più presto la pace e che bisogna stare attenti a

Avanzare semplici dubbi sul fatto che sui vaccini occorresse una maggiore farmacovigilanza, come più volte questo partito ha messo in evidenza, era tutelare la libertà, sì o no? Lo era, anche alla luce dei fatti che sono venuti fuori oggi, che testimoniano proprio che ci sono stati effetti avversi e lo stanno dicendo in tutto il mondo *(Applausi),* compreso il famoso Fauci,

Cartesio diceva che il dubbio è all'origine della conoscenza. Allora, la domanda che facciamo è la seguente: bisogna difendere la libertà sempre e comunque, non va difesa solo dal fascismo, dal comunismo e da tutte le forme di autocrazia, ma si difende sempre e comunque. Su questo noi ci saremo, altrimenti il sacrificio di Giacomo Matteotti sarà risultato

procedura d'urgenza. Voglio ringraziare i rappresentanti di tutti i Gruppi per il sostegno convinto, che oggi viene testimoniato da tutte le loro adesioni, in particolare quella del presidente della Commissione cultura Marti. Questo disegno di legge ha tra i firmatari i nomi di tutti i senatori a vita e, tra essi, come prima firmataria Liliana Segre. *(Applausi)*. C'è un passaggio in particolare del suo discorso inaugurale, che tenne qui in Senato il primo giorno della nuova legislatura, che oggi voglio citare: «In Italia il principale ancoraggio attorno al quale deve manifestarsi l'unità del nostro popolo è la Costituzione repubblicana che - come disse Piero Calamandrei - non è un pezzo di carta, ma il testamento di 100.000 morti caduti nella lunga lotta *(Applausi)* una lotta che non inizia nel settembre del 1943, ma che vede idealmente come capofila Giacomo Matteotti». Giacomo Matteotti e il coraggio e la lucidità che ebbe nel denunciare la natura strutturalmente criminale del fascismo sono alla base della riscossa che venne poi, che è a fondamento della nostra Repubblica. Matteotti venne ucciso perché la sua condanna del fascismo, nel discorso del 30 maggio del 1924, fu circostanziata e implacabile. Fu l'atto di accusa contro i brogli elettorali e la violenza squadrista che ovunque, nelle elezioni del 6 aprile (quelle dell'antidemocratica legge Acerbo), aveva impedito ai candidati delle opposizioni di svolgere comizi, affiggere manifesti o andare a votare: una violenza brutale e bestiale che fu da sempre strumento del fascismo, lo squadrismo contro ogni oppositore e in particolare contro i socialisti, con le devastazioni delle Case del popolo, delle Camere del lavoro e delle tipografie con l'assalto alle case private, nelle città e nelle campagne. Matteotti aveva denunciato tutto questo, dall'inizio, senza tergiversare, sfidando il fascismo e Mussolini a viso aperto. Già nel 1922 aveva pubblicato un'inchiesta sulle violenze dello squadrismo fascista e nell'aprile del 1924, nonostante gli fosse stato requisito il passaporto, era stato a Londra con il Labour party e fu il primo a denunciare in Europa il pericolo assoluto del totalitarismo fascista. Il 30 maggio intervenne alla Camera e l'eco fu enorme. Pochi giorni dopo, il 10 giugno, venne rapito e ucciso dai sicari della polizia fascista, per volontà di Mussolini, che ne rivendicò poi la responsabilità il 3 gennaio dell'anno successivo, instaurando a tutti gli effetti, senza più finzioni, il regime dittatoriale. Mussolini volle la morte di Matteotti, spaventato dalla sua tenacia di oppositore e dalle sue indagini sulla corruzione del Governo e della cerchia dello stesso Mussolini. Il fascismo è stato una dittatura fondata sull'omicidio del deputato Giacomo Matteotti e per questo - come ha scritto il presidente Mattarella - non può esserci oblio, perché la Resistenza e la Liberazione hanno le proprie radici nella testimonianza di personalità come Giacomo Matteotti. *(Applausi)*. Matteotti fu un combattente e un martire della democrazia, che non si piegò mai. Il suo antifascismo fu tutt'uno con la difesa degli ultimi, con la battaglia per i diritti dei lavoratori e con l'impegno per l'emancipazione di contadini e braccianti, a cominciare dal Polesine, la sua terra natale; una lezione attuale, oggi più che mai. Ricordare Matteotti, farlo vivere e prendere esempio da lui è militanza attiva, non di parte, ma cittadinanza che accomuna tutti: la sua figura appartiene alla nostra intera democrazia, a tutta la Repubblica italiana e in qualche modo ne è il simbolo, con il suo eroismo, la sua passione e la sua generosità. Nessuno aveva ordinato a Matteotti di pronunciare quel discorso; anzi, tutte le circostanze, la violenza, l'intimidazione e la chiamata in correità avrebbero indotto a fare l'opposto, a non parlare, ad acconciarsi, ad accomodarsi, a mimetizzarsi ad essere complice. Invece, egli si alzò, in un'Aula come questa, e volle parlare, denunciando il fascismo. Il fascismo non è un'opinione, è un crimine, dirà anni dopo Sandro Pertini *(Applausi)*, che volle iscriversi al Partito socialista, di cui Matteotti era segretario, in seguito alla sua morte e volle che sulla tessera ci fosse la data del 10 giugno, il giorno del suo rapimento e assassinio. Quella data, Presidente, il prossimo anno compirà cento anni, ma non importa quanto tempo sarà passato: è una data viva, perché parla e ammonisce il tempo di oggi; è uno dei tornanti più drammatici della nostra storia e uno dei più significativi per i valori di democrazia, libertà giustizia sociale incarnati dalla nostra Costituzione. Per questo sarà importante - e concludo - costruire intorno a questa data una pedagogia civile e alla figura di Matteotti un senso di appartenenza,

della nostra storia e di consegnare ai più giovani il senso del legame che c'è tra memoria e futuro, un patto condiviso tra le generazioni, un patriottismo repubblicano.

per la quale Matteotti si è battuto a costo della vita, che è un grande Paese, libero e democratico come egli sognava. *(Applausi)*.

Grazie, Presidente. innanzitutto vogliamo annunciare, come Gruppo Fratelli d'Italia, il voto favorevole all'adozione della procedura abbreviata per il disegno di legge sulle celebrazioni del centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, che cadrà il 10 giugno 2024. Conosciamo la storia di Matteotti, ma la ricordiamo. Quando fu ucciso, Matteotti aveva solo trentanove anni, ma alle spalle aveva già un lungo impegno politico, iniziato oltre vent'anni prima e vissuto sicuramente con coraggio e passione. Aveva infatti molto spesso assunto posizioni scomode e difficili. Durante la Prima guerra mondiale, si espresse così fortemente contro la partecipazione dell'Italia al conflitto da essere condannato al confino in Sicilia dal 1916 al 1918. Ricordiamo che, tornato alla politica fin dal 1919, fu tra i più strenui oppositori del fascismo. Nel 1920 e nel 1921, nell'ambito del Partito socialista italiano, si oppose alla fazione comunista, che non aveva ancora dato vita a un partito per conto proprio. Nel 1922, pochi giorni prima della Marcia su Roma, fu espulso dal partito insieme a Filippo Turati, Giuseppe Modigliani, Claudio Treves e altri, tutti accusati di aver partecipato alle consultazioni del Re per la formazione del nuovo Governo. Gli espulsi fondarono il Partito socialista unitario, di cui Matteotti divenne segretario nazionale. Fu eletto deputato nel 1919 e nel 1921. Lo fu anche nelle elezioni dell'aprile del 1924, con la nuova legge elettorale che attribuiva un premio di maggioranza alla lista che risultasse la più votata, a condizione che superasse il 25 per cento dei voti validi. I risultati pubblicati dal Ministero dell'interno attribuirono il 60 per cento dei voti alla Lista nazionale guidata da Benito Mussolini, che includeva non solo candidati fascisti, ma anche parecchi liberali, come Orlando e Salandra, ex popolari, cattolici e tanti altri ancora. Il 30 maggio Giacomo Matteotti intervenne alla Camera dei deputati, affermando che nessun elettore italiano si era trovato libero di decidere con la sua volontà, a causa delle intimidazioni durante la fase di presentazione delle liste, nel corso della campagna elettorale e anche nei seggi. Di conseguenza, affermò che era dubitabile che la Lista nazionale avesse ottenuto quel 25 per cento necessario al premio di maggioranza. Undici giorni dopo, il 10 giugno, giorno nel quale era atteso un suo nuovo intervento alla Camera, uscito dalla sua abitazione sul Lungotevere, venne caricato a forza su un'auto da una squadra di cinque uomini, parte di un gruppo segreto fascista legato al Viminale, che si era scelto il nome di Čeka, quello della polizia politica sovietica. Secondo le ricostruzioni, Matteotti lottò e uno dei sequestratori lo colpì mortalmente con un pugnale. I cinque finirono per seppellire sommariamente il cadavere. Amerigo Dumini, che comandava la squadra, fu arrestato due settimane dopo. Dal punto di vista politico, la vicenda mise per mesi in gravi difficoltà il primo ministro Mussolini, da molti indicato come il mandante, che ne uscì con il discorso alla Camera del 3 gennaio 1925, nel quale affermò di assumersi ogni responsabilità di quanto era avvenuto. Dal punto di vista giudiziario, nel 1926 Dumini e altri due uomini della squadra furono condannati a quattro anni, di cui tre cancellati da un'amnistia, per omicidio preterintenzionale. Nel 1947 si tenne un nuovo processo, in cui Dumini fu condannato all'ergastolo per omicidio premeditato. Sei anni dopo, però, fu scarcerato in virtù dell'amnistia promossa e voluta da Palmiro Togliatti, capo del Partito comunista. L'insegnamento che si deve trarre da questa data, in questa fase storica, in cui i valori di un Paese veramente democratico non possono che essere condivisi, dalla figura e dalla vicenda di Giacomo Matteotti oltre naturalmente al rifiuto, alla condanna della violenza nel confronto politico, da qualunque parte provenga, e all'importanza del rispetto delle regole democratiche, cose che riteniamo tutti scontate, ma che è sempre bene sottolineare e ribadire è quello di difendere sempre il diritto, che per un parlamentare e un esponente politico è anche un dovere, di denunciare le storture, di criticare quanto si ritiene metta in pericolo le istituzioni di esprimere le proprie convinzioni su quale sia il bene della Nazione e delle sue istituzioni. Auspichiamo che tutto questo emerga nello studiare la figura di Giacomo Matteotti nel centenario della sua morte. Presidente, vorrei concludere citando una frase del discorso di Matteotti del 30 maggio 1924. Al Presidente della Camera, che lo invitava a proseguire il suo intervento nonostante le interruzioni dei tanti avversari,

il parlamentare deve sempre parlare come tale, esprimendo le sue convinzioni sugli interessi della Nazione e dei suoi concittadini. Questo è il nostro diritto ed ancor più il nostro dovere. Per questi motivi, ribadisco il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi in discussione, di iniziativa della senatrice Giulia Bongiorno, si inserisce in un percorso che è stato inaugurato dall'approvazione del cosiddetto codice rosso, norma fortemente voluta dalla medesima senatrice, al tempo Ministro della funzione pubblica. È una riforma della normativa esistente, al fine di dare una risposta a fenomeni delittuosi molto gravi di violenza di genere, che purtroppo ancora insistono. Si rammenta, per quanto qui di interesse, che la norma prevista nel codice rosso, la legge n. 69 del 2019, in particolare all'articolo 2, introduce una norma in base alla quale, per una serie di delitti, ricondotti alla violenza di genere e domestica, il pubblico ministero è tenuto ad assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha denunciato i fatti di reato entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della *notitia criminis.*

La direttiva impone agli Stati membri di provvedere affinché l'audizione della vittima si svolga senza indebito ritardo dopo la presentazione della denuncia. Il termine dei tre giorni inserito dal codice rosso è stato considerato ordinatorio già dalle prime applicazioni, vista in realtà l'assenza di una comminatoria di nullità o l'inutilizzabilità dell'atto compiuto oltre il termine. vedere, in realtà, era stata introdotta una sorta di protocollo investigativo di matrice legislativa. È stata effettuata nel frattempo un'analisi di impatto della disciplina;

che alcuni uffici di procura, per esempio, nell'applicazione della deroga prevista dalla legge circa il rispetto del termine dei tre giorni hanno individuato una sorta di casistica dettagliata. Invero, la problematica è che, a volte, il termine dei tre giorni non è stato rispettato. La senatrice Bongiorno insieme ad altri colleghi senatori ha proposto pertanto un disegno di legge finalizzato a superare questo *vulnus*, che è grave perché purtroppo, come emerge anche dalle notizie di cronaca,

assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti entro i detti tre giorni dall'iscrizione della *notitia criminis*. Il testo originario prevedeva che, nel caso in cui il pubblico ministero non rispettasse il termine dei tre giorni, il procuratore generale presso la corte d'appello potesse avocare a sé le medesime

si è giunti invece a proporre un testo che interviene in materia di titolarità dell'azione penale, quindi sul decreto legislativo n. 106 del 2006. 106 del 2006. Nel caso in cui il pm assegnatario dell'indagine non proceda nel termine dei tre giorni all'ascolto della persona offesa, si prevede che il procuratore della Repubblica, titolare esclusivo dell'azione penale, possa revocare l'assegnazione del procedimento, procedendo direttamente o attraverso l'assegnazione ad altro magistrato dell'ufficio per provvedere all'assunzione di dette informazioni, salvo che non emerga la necessità di tutelare minori o la riservatezza delle indagini. Il disegno di legge inoltre, in materia di disciplina di attività di vigilanza da parte del medesimo procuratore generale presso la corte d'appello, prevede che questi sia tenuto ogni tre mesi ad acquisire dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine del termine entro il quale devono essere assunte le informazioni, nonché a inviare al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale, per monitorare l'andamento di dette denunce. Di conseguenza, il testo approvato dalla Commissione ha comportato anche la modifica del titolo. La norma interviene quindi in una materia molto complessa, sulla quale è continuo il confronto al fine di combattere quotidianamente un odioso fenomeno che necessita di continui

Signor Presidente, interverrò brevemente sul disegno di legge in esame solo per dare un contributo conoscitivo. Nel merito delle norme interverrà in modo più puntuale il senatore Zanettin in dichiarazione di voto per il Gruppo Forza Italia. La modifica normativa proposta dalla presidente Bongiorno, che ringrazio, nel testo modificato dalla Commissione giustizia si inquadra nella necessità di rendere più efficaci alcune disposizioni del cosiddetto codice rosso. Ci auguriamo che i tre giorni, ora diventati perentori, per sentire la persona offesa siano sufficienti a salvarla. Purtroppo, a volte, appena il carnefice viene a conoscenza della denuncia, agisce per vendicarsi. Certamente però non lasciare nulla di intentato ci sembra il minimo per favorire una più puntuale attuazione del codice rosso, che è quella di evitare la morte di una donna già vittima di violenza. Purtroppo le fredde statistiche ci dicono che quindici donne uccise ogni cento avevano denunciato il proprio carnefice. Anche la sola idea di poterle salvare tutte e quindici, riuscendo ad acquisire ulteriori informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, ci sembra un risultato ulteriore, che dobbiamo certamente raggiungere. Poiché le donne ammazzate nel 2022 sono state 125, adottando tutti i provvedimenti nei confronti del potenziale omicida avremmo salvato diciotto donne e questo sarebbe già stato un grande risultato,

che non sia solo il 15 per cento delle donne a denunciare, ma che tutte vengano rese consapevoli della necessità di presentare una denuncia contro il proprio aguzzino. sono infatti i reati spia che potrebbero far passare dalle persecuzioni alle violenze e che forniscono anche indicazioni sul passaggio a reati ancora più gravi, fino al femminicidio. Ecco perché va salutato con favore questo ulteriore passaggio normativo. L'augurio è che si proceda a ulteriori tagliandi al codice rosso, che resta una conquista normativa fondamentale da difendere, migliorare e integrare. Serve una maggiore sensibilizzazione nei confronti delle donne, per dotarle di strumenti che le aiutino a valutare senza dubbio i propri aguzzini e a denunciarli, dando alle vittime la certezza che verranno protette. Bisogna fare in modo che quel catalogo di reati che ogni anno ci viene fornito dal Ministero dell'interno, di solito l'8 marzo nella Giornata internazionale della donna, diventi un inventario di azioni positive a favore delle donne.

oggi al nostro esame ha una grande importanza nella strategia del tempo di reazione che il legislatore già in precedenza ha deciso di valorizzare con la norma del cosiddetto codice rosso, quando ci troviamo di fronte a particolari e riprovevoli reati. Il tempo gioca un ruolo importantissimo nella possibilità di garantire un intervento giudiziario efficace sui casi di violenza di genere e su tutti quelli di abuso sessuale in ambito familiare e - come si dice, non tecnicamente - domestico. La strategia che il legislatore in questo caso vuole utilizzare riprende, in maniera forse parallela, quella che si chiama avocazione, anche se in questo caso tecnicamente non lo è.

che prevede, in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero e precisamente all'articolo 2, i poteri che possono essere esercitati dal procuratore nel momento in cui affida incarichi ai magistrati del suo ufficio.

vecchio in ambito giudiziario. Ci troviamo pur sempre di fronte a un presidio costituzionale essenziale per la funzione di salvaguardia del principio di effettività dell'azione penale: ricordo che il pubblico ministero è tenuto all'attuazione oggettiva della legge in ogni momento della sua attività e nell'applicazione di questa legge ha spazi di manovra che sono stati rigorosamente contenuti e circondati da una fitta rete di controlli. Tuttavia, lo strumento dell'avocazione - ed è il motivo per cui si è deciso invece di utilizzare un'altra strategia normativa - ha un semplice problema, che spiegherò ai colleghi. Il numero di procedimenti per i quali periodicamente le procure segnalano condizioni di stallo è tale che, se fosse sistematicamente utilizzato lo strumento dell'avocazione, questa smetterebbe di costituire un'eccezione rispetto al principio per cui è il procuratore della Repubblica il titolare del potere-dovere d'indagine e di azione. Ci dovremmo poi chiedere come muoverci con il Consiglio superiore della magistratura, che addirittura ha approntato un documento su criteri di priorità e gestione dei flussi di affari, di affari, per risolvere il problema dell'impossibilità per gli uffici della procura generale di esercitare massivamente il potere di avocazione. Quando ci troviamo di fronte a reati gravi come quelli che riguardano la sfera familiare, dobbiamo

procedimentale, tale per cui non si riesce a garantire una risposta ai soggetti vulnerabili come le vittime di abusi, che purtroppo sono perlopiù minori e a volte anche donne in stato di gravidanza, che vengono fatti oggetto di condotte riprovevoli in ambito come i maltrattamenti. Ebbene, dovevamo garantire a queste persone una risposta efficace al ritardo del pubblico ministero che, purtroppo, spesso e volentieri non mantiene il termine dei tre giorni stabilito nel codice rosso per audire la persona informata quale condizione indispensabile per conoscere cos'è accaduto tra le mura domestiche. Ci sembra un ritrovato tecnico di assoluta efficacia, perché voglio ricordare che nella previsione che ho citato prima, ovvero l'articolo 2, quando si parla di criteri a cui attenersi da parte del magistrato delegato, può ad esempio anche insorgere, oltre a un mero ritardo, un contrasto tra il procuratore delegante e il magistrato a cui è affidato l'affare. È assolutamente indispensabile che si sviluppi immediatamente una reazione tale da garantire che quel procedimento vada avanti.

la situazione generale e la procura trasmetta quindi informazioni al procuratore generale presso la corte d'appello per fargli sapere in quali e quanti casi il pubblico ministero ha mancato, ad esempio, una notifica di avviso di conclusione delle indagini oppure non si è determinato sull'azione penale. Anche

quanto a profili di tardiva azione dell'inquirente, si possono ovviamente concretizzare anche casi di rilievo deontologico, per omissione nel compimento di attività doverose durante la fase delle indagini preliminari.

dobbiamo affinare quotidianamente gli strumenti in mano agli organi inquirenti e alla polizia, ma anche agli avvocati, alle associazioni e a tutti gli enti che organizzano, ad esempio, i corsi per uomini maltrattanti.

ovvero il riproporsi di nuove situazioni in cui l'autore dei fatti si mette nuovamente

è un fatto positivo, ma ci induce anche a fare grande attenzione a non spostare l'accento, che deve rimanere innanzitutto sulle donne vittime di violenza, sulla loro volontà, sulla difficoltà dei loro percorsi e sul fatto che dovrebbero trovare intorno a loro atteggiamenti di ascolto non giudicanti, ma di sostegno. Lo dico perché nell'insistere sul fatto che ci siano tempi prescrittivi, si finisce per avere invece un tono giudicante.

tornare nuovamente a essere interrogata dal pubblico ministero, viene prima la nostra idea della norma o il rispetto della condizione di quella donna *(Applausi),* che invece ha bisogno di tempo per per ragionare, per pensarci, per consolidare la sua necessità o magari anche per sconfiggere le paure che possono venire dopo una denuncia su cosa sarà il suo futuro e quale sarà il suo avvenire come farà a farcela? Credo che questa domanda dobbiamo farcela, perché ogni tanto sento prevalere l'idea che fare giustizia prescinda dalle vittime

quanto tempo ci mettiamo ad attuare le indagini, quali sono le punizioni o quante risorse diamo da una parte. Se invece Se invece affermiamo, come facciamo quotidianamente - perché credo che su questo siamo tutte e tutti d'accordo - che la violenza maschile contro le donne è un grande tema culturale, oltre che di responsabilità penale ed etica degli uomini che la commettono, se è questo, cioè se è un fatto ormai sistemico, che bisogna contrastare dal punto di vista della cultura, servono norme che non guardino ai singoli aspetti, ma propongano temi generali, e mettano tutti gli strumenti possibili a disposizione

anche una risposta celere per i cittadini e per le cittadine sul terreno della giustizia, ma spesso è più facile che quella risposta di celerità venga da processi di specializzazione, da aumento degli organici e da risorse effettive, anziché semplicemente dal fatto di adottare logiche che, alla fine, diventano punitive, perché non rispettano prescrizioni prescrizioni quotidiane.

Quello che ha detto la collega Camusso inerisce a un tema molto articolato, perfettamente condivisibile, tant'è che la stessa Commissione

tutelare le vittime di violenza. La proposta mira soltanto a procedimentalizzare in misura più efficace la scansione temporale del passaggio dal procuratore della Repubblica al magistrato: ascoltare prima le motivazioni per le quali il magistrato non ha la persona offesa ha anche la finalità di tutelarla. Ci potrebbero essere motivi legati alla sicurezza o alle indagini, quindi l'emendamento è stato proposto al fine di far sì che la vittima sia ascoltata, perché proiettare indirettamente sul procuratore generale la gestione e l'audizione della donna potrebbe lederla nell'evolversi del

sui percorsi riservati agli uomini autori di violenza, cercando anche di fare in modo di intercettarla ai primi segnali. Chi se ne sa che è falsa che è falsa la narrativa del *raptus* per cui improvvisamente, in una coppia in cui tutto andava bene, l'uomo si sveglia la mattina, impazzisce e uccide la compagna. Non succede così, ci sono tantissimi segnali che a volte si manifestano per anni. Lo strumento dei percorsi per uomini maltrattanti, agganciato anche all'ammonimento del questore, può fare in modo che i loro comportamenti vengano intercettati prima che la violenza raggiunga livelli drammatici.

di euro annui dedicato al supporto di questi centri che sono ancora allo stato quasi pionieristico in Italia,

i tradizionali centri antiviolenza che si occupano delle vittime di violenza una volta che è stata subita, ma anche dei centri dedicati agli uomini maltrattanti, che sono quelli che - grazie ai professionisti che vi operano fare in modo che la violenza non raggiunga il suo apice estremo. È stata chiesta una riformulazione dell'ordine del giorno nella quale viene espunta proprio la parte che riguarda i centri per uomini autori di violenza. Per noi questa è una scelta incomprensibile, quindi rilanciamo la formulazione iniziale, chiedendo, se possibile,

Presidente, colleghi, membri del Governo, esistono argomenti - ringrazio il senatore De Poli e la senatrice Biancofiore per avermi permesso di intervenire - che non vorrei mai affrontare, intanto perché si tratta di violenza, poi perché è violenza tendenzialmente o quasi esclusivamente di genere, ma anche perché è correlata a un elemento che in qualche modo è sacro

lo stereotipo della tranquillità, è l'ambiente domestico, una specie di nido morbido, accogliente; purtroppo, però, negli anni, nei secoli e anche stamattina, scopriamo che è pieno di spine,

ma perché evoca in noi un'insicurezza e una perdita di certezza rispetto alla famiglia e all'ambiente domestico. Nelle ore grigie e complicate che in ognuno di noi mordono il cuore e l'anima, essere rassicurati da queste realtà ci serve, ci dà calore all'anima. Purtroppo, la notizia costante di queste violenze

la violenza da sempre; avrei voluto cambiare mestiere, ma è troppo affascinante quello che ho fatto e faccio - ci fa inciampare l'anima. Dobbiamo però porci un punto fermo: certamente la violenza più evidente è la morte della compagna, della moglie o della sorella di un uomo violento;

che ci colpiscono per la loro brutalità più evidente, oserei dire più medica. Questa è la violenza più deprecabile - ci mancherebbe altro - ma non è solo questo. La violenza è il ricatto economico del maschio rispetto alla compagna; è la privazione di una libertà

violenze inaudite, che sembrano invisibili, ma non lo sono e non lo devono essere. Ecco perché sono d'accordo con la senatrice Camusso, dice che gli organismi giudicanti devono continuamente essere aggiornati dal punto di vista culturale, soprattutto in relazione alla personalità femminile, che per fortuna non è uguale a quella maschile, ma che ha enormi potenzialità e qualche volta fragilità, soprattutto nella cultura circostante, che enfatizza i danni che il maschio può produrre. Spendo una parola per qualcosa che spesso non è conosciuta. Chi, come me, ha cercato di studiare per decenni questo straordinario universo che è il bambino ne ha fatto una cultura costante.

non solo perché teme ripercussioni e vendette da parte della persona cosiddetta forte (concluderò su questo), ma perché si colpevolizza. un bambino subisce violenza da un adulto, soprattutto maschio, il danno più forte che riceve è quello di diventare fragile, perché si sente in colpa.

provvedimento legislativo, al quale plaudo, bisognerebbe inserire, nella coscienza cosiddetta collettiva della struttura sociosanitaria del territorio, centri diffusi, interattivi e culturalmente validi di ascolto e di azione, in difesa dei bambini - lo dico per contiguità - e delle donne.

vivere nella donna una maggiore coscienza di sé e dei propri diritti, ma questo meccanismo un po' arcaico,

dell'apparecchiatura che mi permette di parlare, sarò brevissimo). Ho il *bonus* disabilità, me ne approfitto da qualche decennio è come il bollo *handicap*, qualche volta ne abusi un po', che male c'è? Perdi qualcosa e ne assumi un'altra. Io credo che, senza medicalizzare, una maggior presa di posizione dei colleghi psichiatri e psicologi sia necessaria. Lo abbiamo fatto con il mio maestro Bollea e con il mio maestro Basaglia: sono stato molto fortunato.

non ci sarà democrazia. Saremo lì lì per averla, ma non c'è democrazia, anche per una sola donna che soffre per colpa dell'energumeno. Una parola sull'energumeno: questi non è un forte,

Non deve diventare l'eroe negativo, il demonio. È un povero deficiente, che si approfitta di una persona purtroppo poco difesa,

di applicarsi in tutti i modi - anche nel condominio di casa, non solo nell'attività legislativa - per difendere le persone

accanto all'attività legislativa, quella della quale in maniera umile sto cercando di occuparmi, io insieme a voi, è fondamentale: accanto all'attività tecnica, bisogna guardare più da vicino le persone che soffrono. Spesso voltiamo l'occhio dall'altra parte e questo, forse, è il torto peggiore. È iscritta a parlare la senatrice Camusso. contrastare e in qualche modo arginare il dilagante fenomeno criminale della violenza di genere. Più precisamente, il riferimento è al comma 1-*ter* dell'articolo 362 del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 69 del 2019, il cosiddetto codice rosso, che imporrerebbe al pubblico ministero, nel caso in cui si proceda per delitti di violenza domestica o di genere, di assumere, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, informazioni dalla persona offesa. Tale termine tuttavia, come ammette la relazione di accompagnamento al disegno di legge, non sempre viene rispettato. Il provvedimento si propone quindi di assicurare una più piena tutela alla vittima di reati di violenza domestica e di genere, garantendo il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria superiore nel caso di ministero designato. Il codice rosso evoca ed esige tempi di intervento immediati da parte dell'autorità giudiziaria, quando vengono denunciati atti di violenza nei confronti delle donne, i quali tante, troppe volte si materializzano in un'*escalation* che porta non di rado a conseguenze estreme. Voglio esprimere tutta la mia amarezza nel dover ancora una volta prendere atto di come il nostro sistema giudiziario si riveli inadeguato a far fronte a un fenomeno che non conosce soste e che viene costantemente sottovalutato. Sappiamo bene che alla base ci sono questioni culturali profondissime e che, per venirne fuori, non bastano leggi repressive, ma è fondamentale che il sistema giudiziario appronti rimedi efficaci, che funzionino veramente. Affinché non perda di credibilità, lo Stato deve dotarsi di strumenti che raggiungano gli obiettivi per i quali sono stati ideati. In questo caso, tutelare le donne dalla violenza prevaricatrice degli uomini violenti dev'essere una priorità assoluta. È evidente che il sistema previsto dal codice rosso non basta, non basta, perché, anche laddove le misure ivi previste funzionano a dovere, le indagini sono lunghe, spesso si concludono dopo anni e, nel frattempo, le donne sono sprovviste di tutela o tutelate in modo del tutto inadeguato. Secondo l'Istat solo il 10 per cento delle donne che subiscono violenza o atti di persecuzione denunciano i propri aguzzini. Secondo l'associazione Donne in rete contro la violenza (Dire) questa percentuale può essere innalzata sino al 27 per cento. In ogni caso, sono sempre troppo poche. Sembrerebbe che non si riesca a venirne a capo. Abbiamo detto che il problema è culturale e che la sola repressione non basta. È fondamentale dunque investire nella prevenzione e nella formazione di tutti gli operatori coinvolti, a tutti i livelli. È fondamentale investire adeguatamente nei centri antiviolenza, garantendo la copertura omogenea di tutto il territorio nazionale e che a questi, che sono luoghi di libertà delle donne, arrivino i finanziamenti adeguati nei tempi giusti. Questa proposta di legge mette a nudo una criticità del sistema e tenta di risolverla. Noi non possiamo che condividere questo tentativo. Mi permetto anche di fare un espresso un espresso riferimento a una grave vicenda avvenuta a Bologna di recente, ai danni di due donne, che mi ha condotto a presentare un'interrogazione al Ministro della giustizia e che riguarda proprio il caso in cui innanzi a una denuncia per violenza sessuale, le misure previste dal codice rosso non hanno funzionato a dovere. È un eufemismo. Come ho già detto, il rischio che non possiamo correre è che le donne si sentano poco o per niente tutelate dallo Stato e che i violenti percepiscano un senso di impunità per le condotte violente e prevaricatrici operate ai danni delle donne. Non possiamo Non possiamo consentirgli di pensare di poterla fare franca. A dircelo è anche la più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, che evidenzia come in Italia esista ancora un enorme problema di mancato riconoscimento della violenza maschile contro le donne in sede sia civile sia penale. Le conseguenze includono una diffusa inerzia da parte dell'autorità giudiziaria nell'adottare misure a protezione delle donne, dei loro figli e delle loro figlie, una bigenitorialità imposta anche in presenza di violenza, l'assenza di valutazione del rischio e il mancato riconoscimento dei diritti umani delle donne. La cosiddetta riforma Cartabia, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recentemente entrata in vigore, nella parte riguardante il diritto civile menziona le situazioni di violenza contro le donne. Mancano tuttavia strumenti volti a verificare il grado di efficacia delle misure introdotte a fronte di pregiudizi e stereotipi radicati e persistenti. Inoltre non si possono non menzionare le richieste di modifica della normativa penale avanzate da buona parte delle associazioni che hanno evidenziato la criticità della normativa appena entrata in vigore, che amplia le ipotesi di procedibilità procedibilità a querela e impone un criterio di esercizio dell'azione penale che rischia di impattare negativamente sui procedimenti relativi alla violenza maschile sulle donne che continuano a scontare tassi di condanna estremamente bassi. Infine sarebbe ora di introdurre il tema del consenso nella norma che punisce la violenza sessuale, sul quale abbiamo presentato un ordine del giorno. Per tutti questi motivi, ritenendo il provvedimento comunque lacunoso, annuncio il voto di astensione da parte del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra.

morta dopo essere stata picchiata con pugni e calci e abbandonata al gelo per sette ore su una scala davanti all'appartamento dove la coppia conviveva. Sul suo corpo sono state riscontrate molteplici lesioni e diverse fratture. Le condizioni di ipotermia per il freddo hanno portato a una crisi respiratoria e al decesso. Questa dinamica terribile non è l'unico aspetto agghiacciante della vicenda. Come si è appreso dagli organi d'informazione, l'altro elemento inquietante è che Sigrid aveva denunciato per ben cinque volte il suo compagno. Un compagno che, a quanto pare, ha processi in corso e condanne per violenze nei confronti di altre persone. È uno dei casi in cui avrebbe dovuto attivarsi subito il codice rosso,

Alle domande dei giornalisti sul perché, la procura si è trincerata dietro il segreto delle indagini, ma è evidente che si tratta di un caso di mancata applicazione del codice rosso. Sigrid non è stata ascoltata con precedenza per valutare il pericolo nel quale si trovava, e lo stesso succede in tante procure italiane. Addirittura circolano formulari con criteri standardizzati per astenersi dall'obbligo di sentire la persona offesa nei tempi stabiliti. Le statistiche dicono che circa il 15 per cento delle donne uccise dal loro *partner* lo aveva precedentemente denunciato, eppure lo Stato non è stato in grado di tutelarle. Oggi siamo qui per rimediare. Ci apprestiamo a votare un provvedimento che introduce una nuova ipotesi di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale generale nei casi in cui il pubblico ministero non assume, entro il termine di tre giorni, le informazioni dalla persona offesa. Si tratta quindi di un altro tassello nella prevenzione dei femminicidi. È chiaro che la persecuzione dei reati contro le donne riscontra anche tutti i problemi del sistema giudiziario, dalla lunghezza dei processi alla mancanza di personale, ma qui c'è di più: nonostante tante campagne di sensibilizzazione, gli operatori sanitari e di polizia tendono a non credere alle donne e a minimizzare gli episodi di violenza come semplici litigi di coppia. Anche per questo è importante che il Parlamento riprenda il pacchetto di norme elaborato dalle Ministre del precedente Governo, con cui si puntava ad aumentare le forme di tutela per la donna dal momento in cui denuncia. Tra le misure c'erano, ad esempio, l'estensione dell'ammonimento del prefetto e l'introduzione dell'arresto in flagranza a tutti i reati di violenza di genere. Quando una donna denuncia, il meccanismo di protezione deve funzionare. Possiamo anche introdurre nuove leggi, ma se non si applicano nemmeno quelle che già esistono, cosa possiamo sperare di ottenere? Pertanto, monitoriamo bene se il rafforzamento introdotto oggi basterà o se ci vorranno interventi ancora più incisivi. In ogni caso, un primo passo è fatto. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie. Signor Presidente, colleghi, voglio premettere che il voto di Azione e Italia Viva su questo provvedimento sarà favorevole, perché non ci interessano le polemiche e guardiamo ai contenuti. Anche quando si fa un timido passo in avanti, non abbiamo difficoltà a sottolinearlo. Al tempo stesso, però, devo riconoscere che quello che stiamo per approvare oggi è un provvedimento e un testo agrodolce, un bicchiere mezzo vuoto, che i colleghi della maggioranza hanno purtroppo perso l'occasione di colmare;

dei problemi che abbiamo davanti e al grado di condivisione che si è costruito tra maggioranza e opposizione sulla necessità di dare una risposta sistemica e a

Mi soffermo brevemente sulle ragioni che mi portano a questa conclusione. Com'è stato osservato, il disegno di legge in esame si propone di restituire effettività al pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere. L'obbligo in questione è stato introdotto dal codice rosso. In base alla norma originaria, il pubblico ministero è tenuto ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti, entro tre giorni. C'è una direttiva europea che impone di fare questo adempimento senza indebito ritardo, però sappiamo anche che il termine di tre giorni è meramente ordinatorio e quindi molte volte viene disatteso. quindi che la proposta fatta, secondo noi, va nella giusta direzione. Proprio per colmare questo *deficit* di effettività, il provvedimento in esame, nel testo approvato in sede referente dalla Commissione, prevede che, nel caso in cui il pm assegnatario delle indagini non proceda nel termine di tre giorni, il procuratore della Repubblica possa revocargli l'assegnazione del procedimento, procedendo direttamente, o attraverso l'assegnazione ad un altro magistrato dell'ufficio, all'assunzione di informazioni dalla persona offesa, salvo che non emerga la necessità di tutelare i minori o la riservatezza delle indagini. Il disegno di legge prevede inoltre che il procuratore generale presso la corte d'appello acquisisca con cadenza trimestrale dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine, che dovranno poi essere inviati al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Ora, com'è evidente, il testo va senz'altro nella direzione giusta, perché sappiamo tutti che le regole senza una sanzione o un presidio rischiano di non essere rispettate. Metto fra parentesi delle criticità, alcune delle quali sono state evidenziate dalle colleghe del Partito Democratico. Ve n'è anche una di merito: penso in particolare al rischio di allungare e complicare ulteriormente il corso delle indagini, inserendo ulteriori passaggi procedurali, oppure al pericolo, disperdendo le assegnazioni, di disperdere il patrimonio di specializzazione di alcuni investigatori. Lo metto fra parentesi, perché comunque facciamo un passo avanti. Come dicevo, però, si tratta di un passo avanti troppo poco coraggioso, che non tiene conto dell'approccio multidimensionale che il tema della lotta alla violenza di genere dovrebbe sempre avere. Penso non solo al versante penalistico, ma anche a quello culturale e alla necessità di un sostegno economico e sociale alle vittime, ai loro bambini e alle tante realtà come i centri antiviolenza. A tutto questo nel provvedimento non si fa alcun riferimento, non c'è nessun approccio sistemico, non ci sono la capacità e il coraggio di guardare a questa tematica coinvolgendo tutte le forze presenti in Parlamento, provando a fare un provvedimento che abbia un peso reale e concreto nella lotta alla violenza di genere. I fatti recenti che hanno coinvolto Martina Mucci, il pestaggio di Monica Bizaj e della sua amica, la brutale aggressione nel piccolo Comune sardo, fanno parte di un elenco penoso che ci interroga ogni giorno e ci deve spingere, dopo lo sbigottimento, a mettere in campo una risposta altrettanto forte. Questo ci saremmo aspettati, ovvero la capacità, all'interno del provvedimento, di una risposta sistemica, forte e coraggiosa ad un fenomeno intollerabile, che purtroppo riempie le pagine di cronaca dei giornali tutti i giorni. In questa prospettiva, il mio non è un appello generico, ma un riferimento puntuale a una proposta che, insieme alle colleghe Bonetti e Carfagna, abbiamo fatto quando eravamo al Governo, a cui faceva prima riferimento la collega Stefani, che ringrazio. Si tratta di un provvedimento che mi auguro non solo venga calendarizzato in Commissione giustizia, ma abbia una corsia preferenziale. Vi è anche un'altra proposta da parte della collega Valente e delle colleghe del Partito Democratico. Credo che questi provvedimenti debbano essere esaminati nel più breve tempo possibile. Mi permetto di suggerire alcuni punti. Innanzitutto, occorre garantire una sicurezza immediata per le donne che denunciano. Questa è una misura a me particolarmente cara: non si tratta di conculcare la loro libertà, ma è intollerabile che una donna che trova il coraggio di denunciare, immediatamente dopo veda un pericolo ancora più grave per la propria incolumità e per la propria vita, senza che lo Stato intervenga. *(Applausi)*. Al tempo stesso, credo che si debbano rafforzare gli obblighi informativi sui provvedimenti di scarcerazione. Credo che l'introduzione di un'ulteriore specifica ipotesi di fermo, che prescinda dal pericolo di fughe e di flagranza, debba essere presa in considerazione, così come l'applicazione della custodia cautelare in carcere in caso di elusione dei braccialetti elettronici. Penso altresì all'estensione dei casi di applicazione del provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e in generale a un utilizzo più severo delle misure di prevenzione e cautelari; alle provvisionali anticipate per le vittime, per ristorarle dai danni subiti; all'attenzione ai minori quali vittime anch'essi dei fatti di violenza a cui eventualmente assistono. Insomma, colleghi, c'erano i contenuti, la condivisione e oggi anche l'occasione. Se non vogliamo modificare subito il testo che ci apprestiamo a licenziare, procediamo per vie autonome, ma facciamolo nel più breve tempo possibile, assegnando a quelle proposte il binario più accelerato, anche perché credo che i molti fatti di cronaca ai quali assistiamo ogni giorno inermi impongano a questo Parlamento e al Senato della Repubblica di intervenire nel tempo più veloce possibile. Questo ci aspettiamo dalla Commissione giustizia; sappiamo che la presidente Bongiorno è molto sensibile su questo tema, quindi ci aspettiamo una risposta.

Come ricordiamo tutti, il codice rosso è stata un'iniziativa della presidente Bongiorno, cui va riconosciuto il merito e va ascritta tutta l'approvazione di quest'Assemblea, del Parlamento intero, del Paese e delle donne. Certamente alcune norme hanno trovato un'applicazione meno agevole, in particolare il termine di tre giorni per l'assunzione delle informazioni, ed è proprio su questo punto specifico che il

dalle colleghe intervenute prima e anche i casi specifici che sono stati illustrati creano grande angoscia, con tutta la consapevolezza che,

ma probabilmente dati culturali che purtroppo non riusciamo a sradicare in una società che per certi versi è malata e condizionata anche da stereotipi assolutamente inaccettabili. Tuttavia, va detto che il

caro, quello dell'organizzazione giudiziaria, perché spesso quando in quest'Aula parliamo di organizzazione degli uffici giudiziari lo facciamo in termini astratti, poi in realtà quando andiamo a vedere nel concreto, troviamo procure sguarnite, organici

si pone il tema della riorganizzazione degli uffici giudiziari di questo Paese, sappiamo tutti che, se vogliamo avere magistrati e sezioni specializzati, strutture efficienti nella repressione dei reati, abbiamo bisogno di uffici giudiziari di dimensioni adeguate. Gli studi che sono stati fatti dal Consiglio superiore della magistratura e credo anche dal Ministero

dei fascicoli che transitano da un pubblico ministero all'altro senza efficacia, nasce dal fatto di avere magistrati veramente votati al tema, specializzati e capaci, quando ascoltano e assumono informazioni da parte di donne, minori o soggetti fragili, di entrare in empatia e capire di cosa si tratta e qual è il provvedimento da assumere, altrimenti rischiamo di di scrivere norme sulla sabbia. Ho sentito giudizi un po' ingenerosi nei confronti di questo provvedimento da parte di alcuni colleghi. Ho sentito parlare di norma manifesto, ma non penso proprio si possa trattare di questo. È una norma che incide su un tema specifico, anche se, come ho detto, per risolverlo davvero occorrono anche altri interventi di carattere organizzativo. Mi compiaccio con il Governo, ad esempio, perché è stato

a reprimere tanti reati anche in materia di violenza di genere. Ciò detto, non posso che confermare la mia stima per la per la presidente Bongiorno, per la battaglia che sta conducendo su questi temi così delicati, che devono essere sempre più strutturati. L'impegno di Forza Italia, che è un partito vicino alle donne,

Il MoVimento 5 Stelle ha cercato con tutti i mezzi legislativi a disposizione di combattere questa piaga sociale che, con cadenza preoccupante, assurge alle cronache quasi quotidianamente. Molto è stato fatto, ma purtroppo molto è ancora da fare. Nella scorsa legislatura il Parlamento tutto si è reso protagonista dell'approvazione della legge n. 69 del 2019, il cosiddetto codice rosso, proseguendo il percorso di adeguamento della legislazione nazionale ai dettati tracciati dalla Convenzione di Istanbul. Prevenzione dei reati, protezione delle vittime e perseguimento degli autori del reato rappresentano le tre P mediante le quali il legislatore ha inteso esprimere la propria azione politica. In linea generale, tale *corpus* normativo ha rafforzato le tutele processuali delle vittime dei reati violenti, con particolare attenzione verso quelli rientranti nell'ambito della violenza sessuale domestica, ha introdotto alcune nuove fattispecie delittuose e ha

conseguentemente accelerando l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Relativamente a tali aspetti, a fronte di notizie di reato relative ai suindicati delitti, si prevede un obbligo di ascolto, salvo casi tassativamente elencati, della persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato. Il legislatore, per mezzo della norma in parola, ha garantito l'intervento dello Stato quasi contestualmente all'iscrizione della notizia di reato.

Tale norma è stata considerata come una delle più importanti del codice rosso, in quanto, da un lato, può considerarsi quale primo di una serie di interventi volti alla tutela della vittima dal punto di vista psicologico e, dall'altro, svolge anche una funzione preventiva, attenuando il rischio che la violenza possa ripetersi. Unitamente a ciò, al fine di evitare che l'ascolto a così breve termine dall'accadimento possa ingenerare un concreto, reale rischio di ipotesi di vittimizzazione secondaria, prevede deroghe nei casi in cui vi sia un interesse confliggente da parte della persona offesa, ovvero di minori coinvolti, ma anche quando l'ascolto sia di impedimento alle indagini in corso. Prendendo in considerazione proprio quest'ultimo aspetto, diverse procure hanno individuato una casistica dettagliata da far ricadere nell'ambito della disciplina derogatoria rispetto al generale obbligo di ascolto della persona offesa. Tali ragioni possono essere distinte in quattro macroaree: la prima, relativa alla protezione dei minori coinvolti; la seconda, attinente al legame dell'autore del reato con la persona offesa; la terza, afferente al mantenimento del segreto d'indagine e, infine, quella riferita ai casi in cui l'ascolto sia inutile, perché il soggetto è già ristretto ovvero perché la vittima è già presso una struttura protetta. L'obbligo di ascolto della vittima entro tre giorni dalla proposizione della querela è il punto centrale sul quale incide il disegno di legge oggi all'esame dell'Assemblea. Il provvedimento che ci accingiamo a votare di per sé è condivisibile. Anche in questo caso si poteva fare meglio, si poteva fare di più? Secondo me, certamente sì. Il MoVimento 5 Stelle in Commissione giustizia sta conducendo un'opposizione responsabile. Anche su questo testo abbiamo presentato un numero di emendamenti assolutamente contenuto. Avremmo potuto fare come Italia Viva, che ha copiato e incollato il disegno di legge di iniziativa governativa - anche prima citato - presentato nella scorsa legislatura e poi lo ha trasformato in emendamenti che ora ha anche ritirato. Noi, invece, abbiamo fatto un lavoro completamente diverso. Il meccanismo che voi create e che porta alla revoca del fascicolo al magistrato assegnatario qualora non rispetti i tempi di ascolto della persona offesa non ci convince del tutto. Non si può spogliare di un procedimento il magistrato e poi valutarne le motivazioni, anche perché - come già evidenziato prima a proposito dell'emendamento all'articolo 362 del codice di procedura penale già sono presenti condizioni derogatorie rispetto al generale obbligo di ascolto. L'emendamento correttivo lo abbiamo presentato, ma purtroppo non è stato accolto. Ciononostante, il presente disegno di legge rappresenta un ulteriore piccolo tassello - lo sottolineo - verso il completamento della legislazione in materia di contrasto alla violenza sulle donne, che ha come base la legge n. 69 del 2019. Il Gruppo che ho l'onore di rappresentare osteggerà sempre, con tutte le forze che mette a disposizione l'ordinamento giuridico, la violenza nei confronti delle donne. Vorremmo avere l'opportunità, anche da opposizione, di continuare a dare il nostro contributo, anche in considerazione del fatto che abbiamo già più volte avuto la prova che questo Governo ha veramente bisogno dei nostri suggerimenti. Per queste ragioni e con questo auspicio, dichiaro il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

Se una donna denuncia di essere vittima di violenze continue, credo che debba ricevere aiuto immediatamente, credo che non ci sia una persona in quest'Aula che non la pensi come me. Certamente, chi deve dare aiuto deve indagare, ma anche proteggere la donna. Per proteggerla occorre capire la gravità della violenza denunziata ed emettere misure cautelari,

Sono donne che escono dal silenzio e chiedono aiuto, ma non lo ricevono, perché la denunzia resta sulle scrivanie.

Le donne vengono massacrate, senza che nessuno spesso abbia ascoltato dalla loro viva voce cosa hanno subito e cosa stanno subendo. Le donne vengono massacrate, senza che nessuno abbia adottato le misure che avrebbero potuto salvarle.

il codice rosso ed è stato condiviso. Non l'ho voluto chiamare legge Bongiorno: l'ho voluto chiamare «codice rosso» e l'ho condiviso. Io l'ho pensato non quando ero Ministro per la pubblica amministrazione, ma quando ero giovanissima a Palermo e le donne uscivano dal mio studio, andavano a denunciare e poi non tornavano al mio studio e non tornavano nemmeno a casa loro. Già all'epoca dissi che non era possibile, perché, se consigliavo a una donna di andare a denunziare, questo aggravava la sua posizione e lo Stato non l'aiutava, occorreva ripensare il sistema. Abbiamo quindi creato il codice rosso, che serviva esattamente a dare uno *sprint* alle indagini, alle indagini, proprio per fare in modo che una serie di reati denunziati, tra i quali - li sappiamo tutti a memoria - maltrattamento in famiglia, *stalking* e violenza sessuale, avessero un tipo di reazione immediata.

che cosa è successo? Ho sentito qualcuno chiedere: se avete creato il codice rosso e le donne continuano a essere uccise dopo la denunzia, cosa significa? Significa che il codice rosso non funziona?

Questa è la vera risposta e lo sapete tutti. Possiamo anche scrivere - lo posso fare io o l'opposizione, ci sono tante donne che stanno lavorando su questi temi - la legge migliore;

credo che tutti siate andati a convegni e abbiate partecipato alle discussioni in cui si chiedeva perché non venisse applicato il codice rosso. Io mi sono sentita rispondere - credo che qualcuno ora l'abbia citato - che il Parlamento ha scritto «tre giorni»,

Ma voi pensate che una donna che chiede aiuto e dice che sta per essere massacrata ed è quasi morta, ha bisogno di un termine perentorio o possiamo aiutarla dopo un annetto, un annetto e mezzo? C'è bisogno di scriverlo? Ci hanno detto sì: dovete spiegarci se il termine di tre giorni è perentorio. Va bene, adesso ve lo scriviamo. Ed ecco che nasce il codice rosso rafforzato.

sono già pronti per essere incardinati. Affronteremo la materia domani, dopodomani, sempre; e, dopo quelle proposte di legge, ne faremo altre, perché qui non ci si arrende, e io non mi sono arresa di fronte alla disapplicazione del codice rosso. Se il codice rosso prevede che i tre giorni sono importantissimi per salvare delle donne, per salvare loro la vita; se i dati ci dicono che 15 donne su 100 potrebbero essere salvate, la seguente: chi non le sta salvando? È un sistema che non va? È un ingorgo? Cosa succede? Credo che il Parlamento abbia un obbligo,

per fare in modo che il termine previsto sia rispettato. È un provvedimento contro la magistratura? È contro le Forze dell'ordine o contro gli uomini? Dobbiamo dividere uomini e donne? Dobbiamo dire alla sinistra di votare in un modo e noi in un altro? Io non sto risolvendo il problema della violenza sulle donne; la Commissione giustizia non vuole risolverlo, ma esiste una legge che avete votato che ha risolto i problemi del Paese? Le leggi servono a fare passi avanti; il codice rosso lo abbiamo votato tutti, ha dato i suoi frutti. Questo è un modo per colmare una lacuna interpretativa; è un modo per dire no, per dire che le donne non possono aspettare oltre tre giorni. Cerchiamo di votarlo tutti senza dividerci.

toni pacati, seri e rigorosi. Per la parte che attiene al Partito Democratico ci proverò, anche se le sollecitazioni arrivate sono davvero tante, e alcune forse richiederebbero risposte davvero molto radicali.

forse addirittura neanche il titolo corrisponde più al contenuto del testo: si tratta non più di un'avocazione, ma di una revoca dell'assegnazione del fascicolo. È stato detto a più riprese. Io provo semplicemente a ricordare a tutti quanti noi che questa è una prerogativa che spetta, già oggi, a legge vigente, al procuratore capo di un ufficio, che è l'unico titolare dell'azione disciplinare. Quindi, quando un procuratore capo pensa che nel merito il fascicolo non stia andando avanti, per ragioni che ritiene utili, può revocare, richiamare il fascicolo e riassegnarlo. Questo già avviene, grazie a direttive del CSM e a prassi giudiziarie; avviene. La senatrice Bongiorno da ultimo ha detto che con questo testo proviamo in qualche modo a irrigidire, a inasprire e a rendere più cogente una legge che sostanzialmente non ha funzionato come dovrebbe. Mi permetterò poi di dire quali sono le ragioni per cui non ha funzionato, ma, proprio perché credo che la materia sia così credo anche che dobbiamo imparare ad ascoltarci e a dialogare. Peraltro, avendo presieduto la Commissione parlamentare d'inchiesta per tanti anni, sapete che ho fatto di questo proprio uno stile: quindi dialogo e ascolto. E allora voglio provare a seguire il ragionamento di chi ha pensato questo disegno di legge.

è, in qualche modo, legato a come funzionano oggi le procure, a come si muovono, alla disponibilità di risorse umane, di risorse strumentali e di mezzi per poter in qualche modo andare avanti in maniera più spedita. Ma di questo nella discussione di oggi non c'è nessuna traccia;

Ma, qualora avesse pure voluto provare a cambiare, avrebbe dovuto sicuramente agire su altri fronti; evidentemente sceglie di non farlo. Non voglio dire che si tratta di una norma propaganda, ma il sospetto ovviamente resta dentro di me. ovviamente resta dentro di me. Provo ad andare al cuore della questione. Tre temi sostanzialmente vengono ricordati rispetto a questo provvedimento, tre obiettivi che si intende perseguire. Si insiste

denuncia nei successivi tre giorni non se la sente di rivivere il trauma di una violenza, perché sente di farsi ulteriore violenza. Molto spesso l'ascolto, se

contro la sua volontà, perché costretta, rischia in qualche modo di apparire poco credibile, perché non se la sentiva. Arriva con uno stato emotivo molto spesso sicuramente importante. Noi abbiamo provato a dare voce a quelle donne; non a trovare dei capri espiatori, ma a dare voce a quelle donne. Abbiamo ascoltato gli operatori dei centri

una donna oggi non denuncia perché tante volte non viene creduta, perché viene messa in discussione la sua parola, perché viene vittimizzata e resa nuovamente vittima. *(Applausi)*. Il tema quindi non è il tempo. Il tema è la qualità delle nostre indagini, chi le fa, con quale spirito le fa, con quale specializzazione e con quale competenza. Noi continuiamo a dire che queste sono le strade maestre. Capisco che molto spesso questo rischia di apparire forse anche troppo impegnativo. Molto spesso le strade che vengono scelte sono quelle più semplici, ma non necessariamente sono sempre quelle più efficaci. Qualcuno mi ha detto che possiamo anche tutto sommato votare a favore, perché danni non ne fa.

mettere sotto accusa i pubblici ministeri. Io non so se le procure e i pubblici ministeri sono proprio quelli che oggi dovrebbero andare sul banco degli imputati. So per certo che, invece, secondo le indagini della Commissione parlamentare d'inchiesta, procure e pubblici ministeri hanno fatto salti in avanti notevoli in termini di specializzazione. Ne devono fare ancora di più, come li devono fare le Forze

una volta li mettiamo al centro della nostra attenzione gli uomini violenti, che agiscono con violenza nei confronti delle donne? Possiamo avere gli uomini violenti al centro della nostra attenzione? *(Applausi)*. Io resto basita

Mi chiedo e vi chiedo: era la strada maestra? Era la strada più giusta? Era la strada più efficace? Personalmente, io continuo ad avere molti dubbi anche perché il nostro testo, che poi riprendeva in gran parte quello in esame, sostanzialmente prova a fare esattamente ciò che vi ho detto, cioè mettere al centro il comportamento degli uomini maltrattanti, aumentando le misure cautelari. Vogliamo parlare di automatismo e di rigidità? Io imporrei un automatismo: quello dell'utilizzo del braccialetto elettronico, sempre e comunque, quando si emette una misura cautelare. È uno strumento di controllo. Adottiamo più misure cautelari! Ricordo su questo il *referendum*, riguardo alle posizioni in quest'Aula di tutti noi, che voleva esattamente mettere in discussione l'utilizzo delle misure cautelari anche in materia di violenza sessuale. Ricordiamocelo, perché credo che sia doveroso per onestà intellettuale rispetto a tutti noi. Quindi, più misure cautelari, più braccialetto elettronico, più specializzazione e formazione degli operatori. I percorsi degli uomini maltrattanti sono qui stati richiamati, come preziosi e importanti. Ecco: in questo caso nessun automatismo. Lì c'è un recupero che va valutato di caso in caso. Queste sono le misure che dovevamo mettere al centro

né bandierine che in qualche modo portano a dividerci. Abbiamo praticato in quest'Aula, su questa materia, convergenze importanti e assolutamente non scontate. Sono convinta che questo percorso non sarà interrotto. Registriamo con favore il fatto che sia stata messa all'ordine del giorno la discussione dei nostri disegni di legge, che mi risulta domani saranno incardinati. incardinati. Vogliamo guardare con fiducia a questo percorso e quindi, nonostante le tante, tantissime perplessità di merito rispetto alle questioni che abbiamo illustrato, noi continuiamo ad avere fiducia. Per questo, il voto del Partito Democratico sarà di astensione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, in questo mio primo intervento in Aula voglio entrare nella discussione di un tema drammaticamente sempre più attuale, come la violenza sulle donne, con le cautele e il rispetto che sempre si devono alle vittime, ma anche con la ferma consapevolezza che serve ogni azione volta a prevenire e contrastare gli abusi e a creare quella rete di protezione intorno alle donne, per aiutarle ad uscire dalla spirale di abusi e violenze, restituendole a una vita, libere. Ogni anno ci troviamo di fronte alla dolorosa conta delle vittime, con i loro nomi, volti e storie; le vite di donne che tutti, in cuor nostro, pensiamo dovevano essere salvate, perché troppo spesso poi, ricostruendo le vicende, si scopre che dietro a quell'estremo atto di violenza ce ne sono stati infiniti altri, in un crescendo di privazioni, di mortificazioni, di minacce, di violenze fisiche e psicologiche. Sappiamo bene ormai quanto sia importante parlare per far uscire dal chiuso delle mura domestiche la paura che quel fatto privato diventi pubblico quella paura di essere sbagliata, di esserselo meritato in fondo o di non vedere altra prospettiva per se stessa o per i propri figli si trasformi invece in coraggio, coraggio di chiedere aiuto, di denunciare, di dire basta. È importante che le istituzioni ne parlino e lavorino con le nuove generazioni per fornire agli uomini e alle donne di domani gli strumenti per comprendere il rispetto dell'altro, anche quando un rapporto finisce, finisce, e che il dolore per un distacco non ci autorizza mai a pensare di ricondurre l'altro a noi con la forza, perché non è un oggetto, una proprietà della quale possiamo disporre, ma è una persona libera di scegliere per la propria vita. Siamo tutti consapevoli dell'importanza di questo cambiamento culturale che parte dalla conoscenza del fenomeno e dalla capacità di riconoscere i campanelli d'allarme, ma soprattutto di saperli ascoltare. Sappiamo però altrettanto bene quanto sia essenziale che a questo lavoro sulle coscienze siano affiancate efficaci iniziative e azioni per intercettare e fermare quella violenza. Con l'introduzione della legge n. 69 del 2019, il cosiddetto codice rosso, si è intervenuti proprio per affrontare la tutela della donna attraverso una più efficace e tempestiva tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere.

il cosiddetto *revenge porn* o la costrizione al matrimonio, fino ai delitti che causano quelle lesioni permanenti che deformano l'aspetto della donna), il codice rosso è intervenuto con misure specifiche volte ad accelerare il provvedimento per eliminare stasi nello svolgimento delle indagini e accelerare la definizione del provvedimento quando si tratti di delitti connotati da violenza di genere. prevedendo che la comunicazione di notizia di reato da parte della polizia giudiziaria al pubblico ministero fosse immediata, anche sotto forma orale, e con l'introduzione del termine di tre giorni dall'iscrizione della notifica di reato entro il quale il pubblico ministero senta la persona offesa o chi ha presentato denuncia o querela, consapevoli dell'importanza di agire tempestivamente in queste situazioni. Proprio su quest'ultimo aspetto si concentrava la modifica dell'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di evocazione delle indagini, nonché dell'articolo 127 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Il disegno di legge voleva introdurre infatti una nuova ipotesi di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la corte d'appello quando il pubblico ministero, nei casi di delitti di violenza domestica e di genere, non assumesse entro il termine dei tre giorni dall'iscrizione della notifica le informazioni dalla persona offesa. Come ricordato, il termine dei tre giorni per l'ascolto della persona offesa era stato introdotto proprio dal cosiddetto codice rosso e chi conosce il *triage* nei pronto soccorso sa che per per codice rosso si intende un intervento immediato, senza perdere tempo. Questa introduzione era quindi intesa, con i tre giorni, a riservare ai procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere un trattamento preferenziale, connotato, fra le altre, dalla misura della celerità nella valutazione delle denunce, al fine di garantire una tempestiva tutela alle vittime per porle al riparo da eventuali e purtroppo frequenti *escalation* di violenza. Con la modifica che andiamo ad approvare al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, il procuratore della Repubblica potrà, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserverà le disposizioni dell'articolo 362 del codice di procedura penale, non rispettando il termine dei tre giorni. Il codice rosso ha imposto infatti al pubblico ministero di ascoltare la persona offesa o assumere informazioni da chi ha denunciato tali fatti entro tre giorni. Nella prassi tuttavia - ed è emerso molto bene nella discussione che abbiamo svolto oggi in Aula - questo termine non è stato purtroppo molto frequentemente osservato. Il provvedimento in esame si pone, quindi, l'obiettivo di ovviare all'eventuale inerzia del pubblico ministero prevedendo un tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria superiore. A più di tre anni dall'approvazione del codice rosso, penso sia non solo possibile ma anche necessario fare delle considerazioni sulla base dei dati e della casistica che abbiamo sull'applicazione della legge, in termini di denunce, di pendenze e condanne. Questa valutazione ci spinge, come con la modifica che oggi è all'esame dell'Assemblea, a intervenire per rendere ancora più efficace la norma. Il tempo di intervento è spesso dirimente rispetto al fatto che una donna vittima di violenza possa avere o meno un domani. Ecco dunque la necessità di un codice rosso rafforzato. Purtroppo - e torno alla mia considerazione iniziale - ogni anno ci ritroviamo di fronte alla dolorosa conta delle vittime, con i loro nomi e le loro storie. Ringrazio il Governo che lo scorso 25 novembre ha voluto commemorare le storie di ciascuna di esse colorando di rosso e scrivendo i nomi sulla facciata di Palazzo Chigi. Proprio perché abbiamo il dovere di fare di tutto affinché queste vite siano salvate, annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia.

concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere***

di forte rilievo nella storia recente della sinistra politica in Toscana. Sacconi è stato impegnato nel sindacato per molti anni. Alla metà degli anni

l'incarico di segretario provinciale metropolitano fiorentino dello stesso partito, fino a che non è stato eletto nel 1999 nel Parlamento europeo, incarico che gli è stato confermato nelle elezioni del 2004. Di Guido ci sarebbero da dire molte cose. Nel 2014 scrisse un libro di memorie politiche, che ne rispecchia bene la natura, la passione e la grande sensibilità per i problemi sociali ed economici. Si definì un politico controvoglia e questo poteva sembrare, perché in lui la passione per l'approfondimento dei problemi, l'amore per i tempi lunghi nel ponderare e nell'assumere le decisioni erano caratteristiche che saltavano agli occhi e colpivano chi aveva occasione di conoscerlo. Ho avuto la fortuna di poterlo sostenere nelle campagne al Parlamento europeo, molti anni fa, quando ero all'inizio del mio impegno politico e avevo bisogno di imparare tanto da quelli più grandi, saggi e misurati di me. Devo dire di aver trovato in Guido Sacconi, sempre in quelle occasioni, un maestro, una persona in grado di fare da punto di riferimento e di insegnare la buona politica, con la P maiuscola. Dall'impegno sindacale aveva tratto una grandissima passione e attenzione per le questioni sociali del mondo produttivo e del lavoro. Sapeva stare, con intelligenza e con il senso complessivo degli interessi in gioco e degli equilibri in campo, a difesa dei lavoratori, sempre con modernità, con una grande apertura alle innovazioni e con la capacità di costruire, nella militanza politica, senso di squadra e collaborazione. È stato anche protagonista di grandi innovazioni politiche nel suo campo: penso al ruolo che ebbe nell'allargamento dai progressisti alla coalizione dei democratici, alla vigilia delle elezioni regionali del 1995, e poi in Europa. È stato un parlamentare europeo modello, vicino al territorio, ma capace di inserire i problemi del territorio nelle questioni di rilievo continentale, in una legislazione complessa e ad ampio raggio, come quella che si fa...

e che sono convinto faccia provare dolore a tantissime persone, donne e uomini, che hanno creduto nella bella e buona politica, nella politica fatta con buona fede e passione, di cui Guido è stato un grande esempio.

Ci sono stati più di 450 sfollati e, a detta del sindaco di Ravenna, probabilmente nelle prossime ore molte altre persone dovranno essere allontanate dalle loro case. Esprimiamo, anche a nome del MoVimento 5 Stelle, vicinanza in particolare alla vittima che c'è stata in queste ore e il nostro cordoglio

del decreto siccità e in questo momento ci troviamo davanti all'ennesima criticità per eccesso d'acqua e per situazioni che il nostro Paese non riesce ad affrontare in maniera programmatica. Quindi si parla non più di cambiamenti climatici, ma di sconvolgimenti climatici. I giovani di tutto il mondo continuano a manifestare e a chiedere attenzione.

ringrazio per avermi concesso di parlare in merito all'alluvione che sta colpendo l'Emilia-Romagna e in particolare le città di Bologna, di Faenza, di Ravenna e altre comunità in quella zona. Si tratta dell'ennesima tragedia in un Paese fragile, che ha un costante bisogno di interventi di natura idrogeologica che che rendano possibile la difesa dal rischio idraulico. Non c'è solo il cambiamento climatico, che ovviamente preoccupa tutti noi; c'è anche stato un progressivo allentamento degli investimenti nel campo del dissesto. Questo non è il momento della polemica. Ovviamente ci stringiamo attorno a quelle comunità, ringraziamo per il lavoro prezioso della Protezione civile, dei Vigili del fuoco, di tutte le forze impegnate in questo momento per salvare le vite umane, ma anche per contrastare i problemi che si stanno determinando. Per esempio, in alcuni casi ci sono degli sfollati, quindi vorrei anche vorrei anche mettere in luce e ricordare l'azione importante dei sindaci di quelle comunità in queste ore. Come dicevo, non è il tempo della polemica, però

di investimento. Da soli gli enti locali non ce la fanno, da sole le comunità locali non possono risolvere questo tipo di problemi; c'è bisogno di una strategia del Paese.

dell'unità di missione Italia sicura e Casa Italia. Bisogna dare attuazione a quella previsione, non lasciare che resti lettera morta, che rimanga una previsione sulla

non saremmo capaci di dare una risposta costante, ma continueremmo a spendere molto di più e ad avere un sacrificio doloroso e inaccettabile di vite umane. Signor Presidente, io mi rivolgo quindi a lei perché si faccia tramite nei confronti del Governo, affinché quello che noi abbiamo votato e condiviso all'unanimità in quest'Aula (lo hanno fatto anche gli esponenti del MoVimento 5 Stelle che portano una responsabilità enorme nella cancellazione della struttura tecnica di missione Italia sicura)

Signor Presidente, mi associo anche io alle parole pronunciate dai colleghi e lo faccio esprimendo un profondo senso di solidarietà con la nostra gente. Sono emiliano-romagnola e parlo a nome

prima di tutto la mia solidarietà e la mia amicizia ai cittadini colpiti da queste calamità, ai nostri amministratori, di qualunque appartenenza politica essi siano, che stanno combattendo veramente contro una tragica sequenza di eventi. Proprio ieri a Cesena, una delle città vicine alle zone più colpite, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che era in visita, ha affrontato il tema dei cambiamenti climatici per richiamare a sua volta l'attenzione delle istituzioni e della politica sulla grande straordinaria sfida che il mondo e noi dobbiamo vincere, se vogliamo costruire un futuro da lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti. Mi associo a quanto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha detto in quella

vadano a chi sa spendere in progetti come la messa in sicurezza dei territori, la pulitura dei fiumi e tutto quanto occorre per fare in modo che ci sia davvero più sicurezza e ricerca sui cambiamenti climatici. esprimo di nuovo la mia solidarietà all'Emilia-Romagna.

dall'altra parte ci ritroviamo adesso con un'alluvione che sta assediando i nostri territori e le due cose mal si conciliano, come dicono anche gli esperti. Oggi il problema delle alluvioni è dovuto anche al fatto che i terreni sono in siccità e quindi male riescono ad assorbire anche la tanta acqua

che i provvedimenti si chiamino Casa Italia o con altro nome, serve sicuramente oggi più attenzione ai territori, servono oggi maggiori investimenti per il dissesto idrogeologico che abbiamo nel nostro territorio. Abbiamo

tanta attenzione e tanti investimenti, che servono e sono importanti per il nostro Paese.

ad un problema di siccità e di emergenza idrica, adesso ci ritroviamo invece troppa acqua da gestire. Questa è una situazione critica che sicuramente il Governo sta gestendo nel modo più adeguato possibile. Il ministro Salvini, infatti, ha direttamente convocato per domani il tavolo sull'emergenza idrica

ma soprattutto per contrastare il dissesto idrogeologico. Questi sicuramente sono provvedimenti importanti, che vanno a tutela del territorio e della popolazione. la nostra vicinanza alla popolazione e ringrazio tutte le Forze dell'ordine e la Protezione civile che sono, come sempre, in campo per la nostra sicurezza e per aiutarci nelle emergenze come